Onorevoli colleghi, giovedì 28 maggio è scomparso Giorgio Albertazzi, uno dei più grandi protagonisti della cultura, del teatro, dell'arte del nostro Paese. Abbiamo perso un autore, un regista, un attore versatile, capace di attraversare con eleganza decenni di storia dello spettacolo e di coniugare tradizione e modernità. Inizia a interessarsi alla recitazione all'indomani del Secondo conflitto mondiale, dopo aver scontato una condanna di due anni per collaborazionismo, per la sua adesione alla Repubblica sociale italiana. Debutta a teatro nel 1949 con «Troilo e Cressida» di Shakespeare, per la regia di Luchino Visconti. Da lì inizia un'incredibile carriera, che lo porta ad essere interprete di alcuni sceneggiati tra i più famosi della nostra televisione; basti ricordare il leggendario «Jekyll» del 1969, di cui fu anche regista, e pellicole indimenticabili come «L'anno scorso a Marienbad» di Resnais, che lo consacrano in pochissimi anni come una celebrità. È stato però il teatro il suo più grande amore, la dimensione e il luogo che erano più congeniali alla sua personalità straripante. È quasi impossibile richiamare i tanti ruoli, classici e moderni, che ha affrontato sul palcoscenico, ma voglio ricordarne due che forse più degli altri raccontano l'unicità dell'Albertazzi attore. Mi riferisco in primo luogo al suo «Amleto», quello del 1964, diretto da Franco Zeffirelli. Per due mesi incantò il pubblico londinese del teatro Old Vic, in occasione del quattrocentesimo anniversario della nascita di Shakespeare, successo che lo portò a essere l'unico attore non di lingua inglese celebrato con una foto nella galleria dei grandi interpreti shakespeariani del Royal National Theatre. L'altro suo grande capolavoro è la trasposizione teatrale di «Memorie di Adriano», libro di Marguerite Yourcenar. Nelle centinaia di repliche, il confine tra il personaggio immaginato dall'autrice e quello vissuto da Albertazzi si è dissolto in un'interpretazione unica e magistrale di un uomo che, ormai anziano, riflette sulla sua vita, i successi, l'amore, la morte imminente, la fine dell'impero. Consentitemi una nota di carattere personale. Ho visto Giorgio Albertazzi molte volte in teatro, apprezzando la sua capacità di andare oltre la recitazione, di essere più che di rappresentare il personaggio che portava in scena. Proprio questa sua dote lo ha reso uno dei più grandi attori italiani del Novecento. Non si limitava al palcoscenico, però, questa sua dote. Ho avuto il privilegio di ascoltarlo raccontare gli episodi più intensi della sua vita ogni volta, è stato profondamente emozionante. Allo stesso tempo ciò che in una personalità così forte mi ha stupito era la curiosità costante sulle vite e sulle esperienze altrui. Giorgio Albertazzi ha vissuto una vita libera, controcorrente, provocatoria, ha accarezzato l'idea romantica di poter morire sul palcoscenico, inseguendo quello che egli stesso considerava il fine della sua vita: quella bellezza che lui sosteneva essere «l'armonia delle imperfezioni». Nel rappresentare la commossa partecipazione del Senato della Repubblica al cordoglio per la scomparsa di questo straordinario artista, invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

Uomo dal multiforme ingegno, Giorgio Albertazzi ha lasciato un segno, uno stigma nell'arte, nello spettacolo, nella cultura italiana ed europea; personalità forte e ingombrante, un passato che gli pesava e gli veniva fatto pesare: la militanza nella Repubblica di Salò e le accuse di collaborazionismo. Albertazzi non ha mai rinnegato la sua adesione agli ideali fascisti e ai miti dell'epopea fascista, in cui una vasta parte dell'Italia si rivedeva e sperava, al di là degli esiti e del giudizio della storia. L'anarchico che era in lui, lo spirito ribelle che ne informava l'azione, l'ateismo che costituiva la sua antropologia ce lo indicavano piuttosto come uomo inquieto, permanentemente alla ricerca del sublime vitale, dell'idea di bellezza compiuta, ma sempre provvisoria, di animale da palcoscenico e della ribalta a cui dedicava se stesso con impegno maniacale, curando il tutto e il dettaglio. Semiologo a suo modo, lui stesso era oggetto di studi semiologici: l'essere ingombrante di per sé significa, di per sé lascia segni, incide nella coscienza collettiva, al teatro come sul *set* cinematografico, negli studi di posa e televisivi, nelle arene e in piazza.

«Amleto», per citare alcune delle sue interpreazioni memorabili e intelligenti regie. È stato anche formatore, *coach* di generazioni folgorate dal suo talento e dalla vivida recitazione dei classici, come pure dei contemporanei. Ai giovani attori ha dedicato energie e consegnato il messaggio della grandezza dei testi, delle letture, dei drammi e delle tragedie. Ha accompagnato la nascita e l'evoluzione del linguaggio, dei ritmi, delle scansioni temporo-spaziali della TV in Italia; il bianco e il nero del piccolo schermo come metafora della Nazione che faticosamente veniva fuori dagli anni bui del Secondo conflitto mondiale e della guerra civile; l'etere che un condensatore contenuto nella scatola magica, posta al centro di tinelli e salotti delle nostre modeste case, avvolgeva il nostro sogno di progresso. Albertazzi aveva il volto di questo percorso onirico, poi mutatosi in *boom* economico e benessere sociale diffuso; mirabilia connesse a monumentali nomi come Dante, Dostoevskij, Tolstoj, ma anche Van Dine con il suo Philo Vance e Stevenson nel dottor Jekyll. Albertazzi ha contribuito a forgiare culturalmente generazioni di italiani avvicinandole al sublime, all'arte, al duraturo. Oggi parleremmo di usato sicuro, di ciò che non tradisce, che è autentico. Nella vita di Giorgio tutti abbiamo intravisto l'ancoraggio, la banchina che finalmente appare nel porto delle nebbie. Spegnendosi il 28 maggio scorso nella casa nella Maremma, è come se avessimo spinto noi tutti il tasto del televisore, consegnandoci inevitabilmente - armi e bagagli - al pulsante del telecomando:

Avremmo voluto vederlo su uno scranno a Palazzo Madama: sarebbe stato impareggiabile senatore a vita di un Senato corroborato dalla sua forte personalità, dal suo incommensurabile talento, dalla sua unicità a interpretare la complessità della vita, la contemporaneità tragicomica. Nell'estate del 2013, quando vennero nominati i nuovi senatori a vita, speravamo fermamente nell'attribuzione del laticlavio a Giorgio Albertazzi. Ora che non c'è più, le istituzioni tutte si inchinino alla maestosità del suo genio e l'Italia renda omaggio al grande artista. *(Applausi).*

ritrovando una coincidenza esistenziale con quell'imperatore alla fine dei suoi giorni. Albertazzi pativa molto la fine della bellezza che si consumava col passare dell'età, il momento in cui l'armonia tra corpo e anima si dissolve con la

Era attore anche nella sua vita privata, seduttore di qualsiasi tipo di pubblico, in scena e fuori. Nato a Fiesole nel 1923, figlio di operai, raccontava di avere recitato fin da bambino a scuola per amore di una professoressa; quindi, con l'adesione a una filodrammatica, si ebbe l'inizio della sua passione, della sua carriera; carriera che iniziò veramente solo nel dopoguerra, superato il triste episodio che lo vide aderire alla Repubblica di Salò nel 1943: iniziativa mai rinnegata e vista come gesto di un ragazzo ventenne patriottico che si illudeva nella possibilità di una rivoluzione sociale e che tra l'altro, nel 1945, gli costò l'arresto e una condanna per collaborazionismo

anche se poi in realtà è stato sempre un uomo libero, forte delle sue capacità professionali. Dopo un inizio un po' in sordina, il salto vero avvenne quando nel 1956 iniziò a fare coppia con la sua Anna, anche sua compagna di vita, riuscendo per quasi un ventennio a essere tra i protagonisti della vita teatrale, proponendo classici moderni, da D'Annunzio a Pirandello, ma anche autori contemporanei

dopo il terremoto di L'Aquila, recitò Dante tra le macerie, convinto che oltre al corpo bisogna dare conforto all'anima.

di romanzi per la televisione e l'autore teatrale. Diceva inoltre: «Alcuni amici sostengono che il mio vero mestiere è l'attore. Altri dicono che avrei dovuto solamente scrivere. Altri ancora che non dovrei mai più fare il regista teatrale. Chissà quali sono fra questi gli amici veramente autentici?». Ci uniamo ai tanti che lo piangono come uno dei massimi esponenti del teatro italiano di tutti i tempi.

Giorgio Albertazzi è stato il teatro, quello che anch'io ho conosciuto da giovanissimo, quando la prosa era un appuntamento fisso della RAI. Ci ha lasciato così, a novantadue anni, uno degli ultimi testimoni di un'epoca forse irripetibile nella storia della cultura e della nostra Repubblica. È stato uno dei grandi interpreti, forse il più grande, che negli anni resero il teatro italiano uno dei più importanti del mondo. Era curioso e versatile - così ci viene raccontato - e sul palcoscenico in grado di frequentare con dimestichezza i classici, da Pirandello a Shakespeare, ma anche attento a tutto quel che di nuovo spuntava in quella fase di massimo fermento in tutto l'Occidente. Sempre pronto a osare, sempre tentato dal gusto della provocazione, dallo spiazzare dallo spiazzare critici e spettatori, portò sul palcoscenico Sartre e Camus, ma anche Moravia e Calvino, con quelle edizioni americane che amava proprio per la loro leggerezza. Mise in scena negli anni Sessanta Arthur Miller e Vitaliano Brancati, con uno dei testi per l'epoca più audaci, «La governante», che parlava di omosessualità femminile e per questo fu vietato dalla censura rigida e sessuofoba di quei tempi. Ancora pochi anni fa, nel 2009, scelse di declamare la Divina Commedia nel teatro di una città, L'Aquila, colpita da un terremoto così straziante per tutto il Paese. Con l'Italia occhiuta e codina Albertazzi non aveva nulla a che spartire; in compenso dimostrava che sotto quel velo polveroso e sottile c'era un'altra Italia vivacissima, creativa, all'avanguardia. In quegli anni, quelli della televisione che funzionava, Albertazzi fece la sua parte portando sul piccolo schermo numerosi capolavori della letteratura classica, sino a un'eccezionale versione de «Lo strano caso del che credo un'intera generazione ancora ricordi. In quella parte che Albertazzi interpretava in modo esemplare, proprio perché rinunciava quasi completamente a ogni sorta di effetti speciali, affidandosi solo alla recitazione, c'è chi ha voluto vedere un riferimento alla sua biografia, il riferimento alla adesione nel 1943 alla Repubblica di Salò, per la quale per la quale ha pagato direttamente in prima persona e che in questi giorni è stata spesso rinfacciata alla sua memoria come una macchia indelebile. Albertazzi fece allora una scelta sbagliata credo che lo sapesse benissimo da solo, ma non per questo non rappresenta un grande uomo di cultura del nostro Paese e della nostra Repubblica. Quando dopo due anni di detenzione uscì dal carcere, non si dichiarò mai fascista e non diede mai segnali di nostalgia per quel regime. Quando il Movimento Sociale di Almirante gli offrì una candidatura la rifiutò. Ma neppure rinnegò mai quella scelta, perché sapeva che era stata dettata non da motivi ignobili,

e lo facciamo con grande rispetto, perché è stato un uomo che ha segnato in positivo l'evolversi della cultura italiana.

nel mio paese quando ero sindaco. E poi mi diede la possibilità e il piacere di avere un colloquio privato con lui. In quell'occasione riuscii a capire di aver a che fare con un uomo straordinario che sprizzava umanità e genialità da tutti i pori. Il ricordo di Giorgio Albertazzi è quello di una personalità artistica eclettica, rivoluzionaria e mai banale. un uomo che esprimeva appieno la propria personalità sul palcoscenico, davanti a un pubblico che sapeva ogni volta entusiasmare ed emozionare. Ha vissuto nella continua ricerca dell'innovazione artistica e della multiformità dell'espressione teatrale. Era un artista della comunicazione e dell'interpretazione, ma anche uno dei pionieri che scoprirono le potenzialità del nuovo mezzo di comunicazione televisivo. Contribuì notevolmente a lanciare negli anni Sessanta la televisione con

Albertazzi è stato tra i protagonisti assoluti della vita teatrale italiana - il suo amore è stato il teatro - e rimarrà nella storia e nei cuori di tutti i suoi numerosissimi spettatori; un artista che non si è mai risparmiato, per passione e per amore di quel suo pubblico che lo ha accompagnato già dal 1956, ne «Il seduttore» di Diego Fabbri, in cui comincia a far coppia con Anna Proclemer, anche sua compagna di vita. Albertazzi

Allo stesso tempo, Shakespeare, Adriano e Dante sono stati una costante ragione di vita: lo spettacolo «Memorie di Adriano» rappresenta il filo conduttore dei suoi ultimi trenta anni di carriera, quando durante ogni interpretazione dell'imperatore raccontava anche un po' di se stesso, di come potesse sentire sue molte delle espressioni e delle battute dello spettacolo. E il suo Adriano raggiunse le 800 repliche. Nel 2004 fece storia il suo Dante dalla Torre degli Asinelli di Bologna, davanti a 22.000 persone. Nel cuore di Albertazzi c'è sempre stato Shakespeare, al punto che - lo diceva lei, signor Presidente - nel 1964, in occasione dei quattrocento anni dalla nascita del Bardo, l'attore ha debuttato al teatro Old Vic di Londra in «Amleto», con la regia di Franco Zeffìrelli, ottenendo di entrare con una foto una foto nella galleria dei grandi interpreti shakespeariani del Royal National Theatre, unico attore non di lingua inglese. È stato un uomo che ha vissuto molto in superficie senza mai essere, in realtà, un superficiale;

Signor Presidente, è difficile descrivere la figura poliedrica e complessa di Giorgio Albertazzi. Attore teatrale, regista, anche cinematografico, scrittore in un'epoca in cui gli intellettuali rappresentavano ancora la voce critica di questo Paese, Albertazzi è il simbolo di un'Italia che ha saputo dare vita a a un'eccezionale stagione di grandi protagonisti nel mondo dello spettacolo e della cultura, anche a livello internazionale. Albertazzi, conosciuto anche come re Giorgio, il vero re Giorgio, degno di essere appellato così, o come maestro, come spesso veniva chiamato, però un personaggio ingombrante, perché - com'è già stato detto da altri oratori che mi hanno preceduta la sua vita si compone di molte luci, ma anche di ombre pesanti e - com'è stato testé ricordato - quella più pesante è sicuramente la sua militanza giovanile nella Repubblica sociale, che in molti non gli hanno perdonato, nonché

la vita di Albertazzi è stata impregnata di poesia e di teatro, che forse sono le due sfere nelle quali la sua esistenza seppe esprimersi al meglio. Dario Fo lo definiva un anarchico e, con lui, aveva condiviso un primo ciclo di lezioni-storia per la RAI sul teatro italiano. Era un ciclo dedicato al Seicento, al Settecento e alla commedia dell'arte, e insieme avevano pensato di riproporne un altro. In tal modo, grazie a questo ciclo di lezioni-storia del teatro, erano riusciti a fare entrare il teatro e la cultura teatrale nelle case degli italiani, quando la TV aveva

Di fatto, la TV italiana compie i primi passi insieme a Giorgio Albertazzi, che debutta nel gennaio del 1954 recitando in diretta la tragedia di Shakespeare «Romeo e Giulietta», nel suo programma televisivo «La prosa del venerdì». L'anno successivo inaugura la trasmissione «Appuntamento con la novella»: un appuntamento che divenne fisso nella TV italiana. Nel 1959 è il principe Myskin nell'opera «L'idiota» di Dostoevskij, diretto da Giacomo Vaccari. Poi è protagonista de «L'anno scorso a Marienbad» nel 1961. E questo solo per ricordare una carriera lunghissima, che lo ha visto impegnato anche in una regia non del tutto convenzionale de «Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde» di Stevenson, fino ad arrivare alla consacrazione internazionale al Royal National Theatre di Londra. E, poi, ancora, lo abbiamo ritrovato in TV con un grande classico della nostra letteratura italiana: lo abbiamo visto cimentarsi in Dante. Albertazzi, quindi, ha dato voce e vita soprattutto - perché il teatro è vita - ai grandi classici della letteratura nazionale e internazionale. In oltre cinquant'anni di carriera Albertazzi è stato un punto di riferimento per intere generazioni di attori e registi, e nel 1994 ha fondato e diretto un laboratorio di arti sceniche.

vari Paesi. Vogliamo concludere questo ricordo con un auspicio e un appello. Pare che sia in arrivo, in un futuro molto prossimo,

la figura dell'artista Giorgio Albertazzi sia adeguatamente commemorata, magari rivedendo qualche punto critico della riforma del 2015 e guardando anche al futuro, per fare in modo che un aspetto così importante della vita culturale e sociale di una collettività possa essere adeguatamente celebrato, sostenuto,

Signor Presidente, credo che il Senato abbia fatto bene oggi a ricordare Giorgio Albertazzi. Non faccio parte di coloro che si lamentano del mancato laticlavio. Ogni qualvolta una grande personalità

a volte, è stato concesso a personalità meno radicate nel sentimento e nella coscienza popolare. Giorno Albertazzi ha avuto anche un'interazione con la politica. Ho sentito

anche un po' autobiografica. Vederlo recitare a Tivoli, come sarà successo a tanti di noi, in mezzo alle vestigia dell'antichità ha creato tante volte una piena suggestione e identificazione tra l'attore e le pagine della storia e delle memorie dell'antica romanità. Per quanto riguarda l'interazione con la politica, Giorgio Albertazzi è stato spesso citato per tutta la discussione sul passato, che non è certo questa l'occasione per riaprire. riaprire. Come hanno ricordato anche alcuni intellettuali e storici, egli aveva fatto della sua esperienza giovanile non un fatto ideologico, ma quasi una scelta istintiva di una generazione in un momento drammatico di scontro e guerra civile per l'Italia. Tale vicenda è stata spesso reinterpretata

perché incasellare in maniera banale Giorgio Albertazzi sarebbe fare un grave torto alla sua memoria. Visconti, Zeffirelli e tante altre personalità hanno incrociato il suo percorso, dal teatro alla cultura popolare, attraverso la televisione. Ricordiamo anche le «Memorie di Adriano» e il fatto che fu un grande italiano,

non è stato solo un grande artista e intellettuale, ma anche una persona che ha curato sempre il modo di essere in scena e la preparazione dei suoi allievi, con un'alta scuola di cultura. Si tratta di un grande interprete della storia italiana, dell'alta cultura, che le istituzioni devono ricordare e che la cultura italiana certamente porterà come uno dei suoi simboli

ipercritico e intelligentissimo, appassionato polemista: un grande artista, di cui l'Italia può andare fiera. Una personalità artistica poliedrica, che cominciò con i fotoromanzi, per passare agli sceneggiati televisivi, di cui molti colleghi hanno parlato, al teatro - naturalmente - al cinema - anche se non troppo - fino ai varietà popolari e televisivi. Egli non evitava di andare anche agli spettacoli di varietà,

con tutte le nuove forme di spettacolo, naturalmente anche con quelle televisive, era una delle sue caratteristiche. Fu un uomo modernissimo, da questo punto di vista, un uomo di scena e di palcoscenico: senza senza il teatro non avrebbe potuto vivere. Il teatro è stato il centro della sua esistenza, di grande innamorato della vita, anche delle donne, del palcoscenico e del suo pubblico. Un uomo che si caratterizzava perché era bello: bella voce, bella presenza, una dizione perfetta, una grande cultura (recitava Dante a memoria, lo sappiamo), una passione per il teatro che molto presto lo trasformò in un divo oltre che in un grandissimo attore. L'amore per il palcoscenico nasce in un teatrino del Cinquecento sopra Firenze dove, ancora studente del liceo «Michelangelo», qualcuno lo invitò a recitare. E poi stava nella villa di Bernard Berenson, il grande critico d'arte, e lì, nella villa «I Tatti», che oggi ospita l'Università europea, cominciò ad osservare il grande mondo che passava da quella villa internazionale; una villa dove il giovane Albertazzi scrutava da lontano, affascinato, i grandi personaggi che vi passavano.

del fascino che il fascismo esercitò su di lui, travolto dalla propaganda di quegli intellettuali, a partire da D'Annunzio, che tracciarono l'ideologia di quel movimento politico. Il ventenne Albertazzi ne fu coinvolto e pagò anche

nonostante avesse questa sorta di matrice che di fatto ha sempre mantenuto, ha operato altre scelte particolari. Ricordiamolo: è stato compagno di strada dei radicali nelle battaglie per l'aborto e per il divorzio, poi candidato alle politiche con il centrodestra nel 1996

che ricordiamo. Voglio poi ricordare Luchino Visconti. Albertazzi partì con lui al Maggio musicale fiorentino nel 1949, l'avete già detto, e questo fu l'inizio e anche il modo di interpretare il teatro perché un incontro con

spesso capita ai grandi fiorentini e non importa citarli. Adesso, ancora vivente, c'è Zeffirelli con il quale faremo un grande progetto

non rappresenta soltanto un'evasione, ma è, come deve essere, una necessità. Che "La Pergola" sia risorta così presto è un segno di grande vitalità dei fiorentini. È come se avessero detto: "prima il teatro". E questo vuol dire moltissimo, vuol dire che il teatro è l'uomo. Ecco perché resiste a tutto, non soltanto alle altre forme di spettacolo come il cinema e la televisione (...), ma anche alle guerre, alle grandi calamità, ai cattivi attori, ai pessimi autori, alle sovvenzioni e alla tecnocrazia. Perciò riaprire «La Pergola», per noi fiorentini, non è soltanto un altro atto della ricostruzione della città, ma è soprattutto un modo per affermare che, malgrado tutto, ci siamo anche noi, vivi e vegeti, a dire la nostra». Vorrei concludere con

«Per lui recitare era la vita stessa, una sorta di medicina necessaria. Entrava in scena e il suo viso, la postura del corpo, la voce cambiavano, mostrando una forza che pareva impossibile dietro le quinte. Per me è stato il simbolo di quell'attenzione costante che ogni uomo del nostro tempo dovrebbe avere per il futuro del teatro. E per la sua necessità nella nostra vita. In questo egli era moderno. Moderno per la libertà, per l'entusiasmo e la curiosità, che lo rendevano giovane, anzi, senza età». Concludendo, rispondo alla collega Montevecchi del Movimento 5 Stelle, che chiede che il nostro migliore omaggio possa essere quello di portare il prima possibile in quest'Assemblea la nuova legge sullo spettacolo. Sono molto d'accordo su questo. Il Governo la sta predisponendo. Presto arriverà

un uomo importante, che ha lasciato un segno in questo Paese, Giorgio Albertazzi. E mi è capitato anche di ricordare delle persone che magari non ho conosciuto o ho conosciuto solamente in parte Oggi, invece, sono a ricordare un amico, un politico italiano, un parlamentare. E tocca ancora a me, signor Presidente, per un motivo molto semplice. Perché l'ho conosciuto alla Camera dei deputati nella XVI legislatura insieme ad altri colleghi. Sto parlando di Gianluca Buonanno, signor Presidente, un parlamentare, un amico, un papà, che ci lasciato un vuoto immenso domenica pomeriggio,

intervento di questo tipo. Forse perché le parole sarebbero state tante, talmente tante da non riuscire a condensarle in un breve ricordo. Ma domenica, signor Presidente, un *tam tam* anche sui *social media* (strumento che, tra l'altro, Gianluca utilizzava con una certa frequenza)

Gianluca, ti abbiamo conosciuto i primi giorni della XVI legislatura e da subito ci siamo detti: ma che tipo questo Buonanno! Spiritoso, pungente, realmente realista. Uomo pratico, ragazzo appassionato, di spirito e molto simpatico; pratica, simpatia e passione che metteva in tutte le cose che faceva, soprattutto quando faceva politica. che ha portato alla ribalta della politica italiana il suo essere, il suo sistema di fare e, viste le migliaia di messaggi di cordoglio e quello che in questi giorni è successo per ricordarlo, direi anche nella vita di tutti i giorni. Un uomo di temperamento, direbbe qualche cronista di pugilato, un uomo veramente con la schiena dritta, un uomo che ha saputo, nelle sue varie e intense

«Gianluca, perché hai due orologi?». La risposta era sempre quella: «Uno di questi due orologi è quello di mio papà: lo indosso per ricordarlo». Questo era il nostro amico, il nostro compagno di molte battaglie. Cinquant'anni, signor Presidente, il bello della vita; un incidente lungo la pedemontana nel pomeriggio di domenica scorsa. Il nostro segretario federale Salvini l'ha ricordato buon viaggio ad una persona leale, coraggiosa, concreta, onesta e generosa, sempre tra la sua gente, sia da sindaco che da parlamentare, da uomo libero e da persona semplice. Un pensiero alla sua compagna - come dicevo prima - e al suo bimbo Nicola. Eppure, signor Presidente - lo dico con grande rammarico a nome di tutto il Gruppo della Lega e non solo qualcuno ha gioito per la sua morte; sui *social network* sono apparse frasi vergognose, degne di persone che non hanno dignità. Provo pena per questi soggetti, signor Presidente; ma tu, Gianluca, non ti curar di loro e nemmeno noi lo faremo. Riposa in pace, amico mio, riposa in pace, amico nostro.

Signor Presidente, anch'io mi associo alle parole di cordoglio appena sentite. Ricordo con grande commozione l'anno scorso, quando, in una trasferta a Berlino per la finale della partita di Coppa dei campioni della Juventus, incontrato lui e suo figlio, un ragazzino delizioso di tredici anni; entrambi accesi e appassionati tifosi juventini. Gianluca Buonanno è sempre stato un parlamentare appassionato: tutti ricordiamo le sue battaglie. È stato un sindaco molto amato, molto vicino a tutti i suoi. Credo, quindi, di poter esprimere il pensiero di tutto il Gruppo di Forza Italia di vicinanza al suo bambino Nicola e alla sua famiglia. *(Applausi)*.

Signor Presidente, capita delle volte nella vita di incontrare persone con cui si litiga sempre, con cui non si è d'accordo su niente, con cui sembra sempre che siamo ad un punto di rottura. Capita, e nella politica capita molto spesso. Buonanno era una di quelle persone con cui penso di aver litigato di più nella mia vita: litigavamo in televisione, litigavamo in Aula alla Camera, non poteva esserci persona più lontana dal mio modo di vedere la vita. Eppure queste litigate, questo modo diverso di pensare, questo suo modo davvero davvero al limite di manifestare le sue idee politiche, anche attraverso esercizi simbolici molto spesso discutibili, nascondevano un uomo fondamentalmente buono. E io così lo voglio ricordare: un avversario politico, una persona con cui non si è d'accordo e con cui era molto difficile andare d'accordo, tuttavia un sindaco, quindi una persona che ha cercato un radicamento nella sua vita, felicissimo di essere parlamentare europeo. L'ultima volta che l'ho visto è stata a Fiumicino. Era felice, sorrideva e diceva: «È un posto meraviglioso, è il mio modo di fare politica, è il mio luogo, niente a che vedere con le istituzioni italiane». Insomma, era un uomo appassionato; si potevano non condividere le sue idee, ma almeno c'era la passione, e questa passione nascondeva bontà (guardando ad altre figure politiche, che magari sono fredde e compassate e nascondono cattiveria). Per questo lo voglio ricordare

Nel ricordo di persone che ci lasciano molto spesso si indulge in enfasi e in amplificazioni di sentimenti e di pensieri a suffragio della sua anima. Mi limito a dire soltanto una cosa, recuperando in parte quanto ha esposto poc'anzi la collega De Biasi. Il senso della passione politica era l'elemento distintivo del collega Buonanno, che ci ha lasciato in modo così cruento e improvviso. Una passione politica che, in modo assolutamente originale, si è espressa espressa anche attraverso gesti, atti e modalità che sono entrati - per così dire - prepotentemente nella cronaca della politica degli ultimi anni. La passione politica è stato il suo tratto distintivo. L'onestà intellettuale e l'impegno profuso con grande coerenza e diligenza credo siano stati la cifra distintiva di un uomo, di un amico, di un parlamentare che deve essere ricordato non perché ci ha lasciato in modo così improvviso, ma perché ha rappresentato un modello originale, che addirittura viene apprezzato e ricordato con rimpianto da parte di di quelli che sono stati i suoi più severi oppositori e che oggi, non certamente per celia, si uniscono agli amici della Lega per esprimere il pensiero di lutto, di costernazione e di vicinanza. Questi pensieri, a nome del Gruppo dei Conservatori

signori membri del Governo, parliamo di una materia che in questo ultimo periodo è diventata particolarmente spinosa per i fatti che si sono verificati in questo primo scorcio del 2016 e che hanno portato alla ribalta della cronaca - come dicevo - fatti gravissimi, perpetrati ai danni di amministratori locali. Questo disegno di legge trae origine, com'è noto, dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la sua attività il 26 febbraio 2015.

Credo sia anche doveroso formulare un ringraziamento sia alla Presidente della Commissione d'inchiesta che a tutti i suoi membri per il pregevole lavoro svolto su questa spinosa materia. Il disegno di legge in esame recepisce quindi gli esiti dell'inchiesta, prospettando alcune modifiche normative in materia penale. Durante l'esame in sede referente sono stati definiti in modo più compiuto tali interventi correttivi. Credo sia anche utile e necessario ricordare che questo testo di legge, che porta la prima firma della senatrice Lo Moro, è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, che hanno aderito

Pertanto, una notevole spinta propulsiva a una rapida approvazione del disegno di legge in esame giunge anche - come dicevo - dall'aumento dei casi di minacce e intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio del 2016. In particolare, ricordo che nelle ultime settimane (gli ultimi atti ai danni degli amministratori locali si sono verificati nella mia isola ai danni di un sindaco uscente lo scorso 4 giugno, la sera prima della votazioni) votazioni) tutti i *media* hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando dal Nord al Sud della penisola. Ricordo altresì che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili - su questo ritornerò anche alla fine del mio intervento e al Parlamento di esaminare e approvare rapidamente la proposta di legge in titolo. Auspico, pertanto, che dopo il proficuo lavoro svolto dalla Commissione Giustizia nell'ambito di un sereno clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione, anche l'Assemblea possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di giustizia e di tutela, portate avanti dagli amministratori locali, che in questo momento si sentono oggettivamente sotto assedio, e alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi. Passando al merito del testo in esame, con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione della evidente portata portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione della integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato), con l'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela qui specificamente considerate e testé richiamate. La proposta originaria del disegno di legge in esame in realtà prevedeva una modifica all'articolo 338 del codice penale, nel senso di prospettare come reato anche la minaccia o le violenze rivolte a singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario; ciò al fine di rendere finalmente applicabile una previsione incriminatrice che fino ad oggi di fatto non lo è stata, proprio perché fino ad oggi si parlava soltanto del corpo politico, amministrativo o giudiziario. Alla luce del dibattito svoltosi in Commissione è stata approvata una modifica ulteriore, nel senso di specificare che costituisce reato anche la minaccia ai singoli componenti di un'autorità pubblica di natura collegiale, quando i medesimi singoli componenti operano al di fuori dell'organismo collegiale. Intervenendo sull'articolo 338 del codice penale, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale, il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Il nuovo impianto normativo consentirebbe di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno a sette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altro mezzo di prova e di raccolta della prova. L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento all'articolo 338 del codice penale - come modificato dalla Commissione in sede referente - tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezza dell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esame introduce l'articolo 339*-bis*

sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. A questo riguardo debbo fare alcune precisazioni. Intanto, in Commissione è stato espunto il riferimento all'articolo 594 del codice il reato di cui a tale articolo (reato d'ingiuria) è stato depenalizzato, quindi è stato espunto dal testo.

sorte delle inesattezze, dei ragionamenti sicuramente non esatti, ho anche presentato un emendamento che ha semplicemente l'intendimento di esplicare meglio il contenuto, a mio parere già estremamente chiaro, dell'articolo 3

taluno si è infatti paventato il timore che l'aggravante possa essere applicata ogni volta che il reato di diffamazione, anche a mezzo stampa, venga consumato ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Infatti, la norma prevede esplicitamente che, perché possa essere applicata l'aggravante prevista dall'articolo 3, è indispensabile che la condotta, anche quella diffamatoria, abbia natura ritorsiva: per fare un esempio pratico, si pensi al giornalista che attui una condotta diffamatoria nei confronti di un amministratore pubblico, che ad esempio abbia ordinato la demolizione della casa di quel giornalista o di un altro soggetto. La natura deve essere quindi assolutamente ritorsiva: si sottolinea che è necessario un *quid pluris* nel comportamento dell'agente rispetto alla condotta contemplata nella diffamazione,

sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. Ma si rimane ovviamente aperti al confronto e alla discussione anche in considerazione di un altro aspetto:

Qualcuno ha sostenuto che si portava la pena per il reato di diffamazione a mezzo stampa, qualora commesso nei fronti di un appartenente a un corpo politico, amministrativo e giudiziario, fino a nove anni.

di tutela estremamente diffusa su tutto il territorio nazionale per i fatti incresciosi che si ripetono ormai settimanalmente. Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non siano amministratori locali, ma aspiranti tali, si è prospettato - con l'articolo 4 del testo in esame - un intervento di modifica dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

c'è ancora la vecchia dicitura in lire - a lire 4.000.000) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative. amministrative. Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento che ci occupa, per dare una risposta concreta all'esigenza di tutela manifestata a seguito - l'ho già sottolineato ma giova ancora ribadirlo degli innumerevoli attentati di cui sono rimaste vittime gli amministratori locali, reputo opportuno invocare un ulteriore intervento del Governo che svolga una funzione di prevenzione e di deterrenza. Mi riferisco alla necessità di un maggiore controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine, da attuarsi - un'esigenza prospettata da moltissimi amministratori locali rimasti coinvolti in questi fatti gravissimi gravissimi - anche con una maggiore diffusione dei sistemi di videosorveglianza. Sappiamo che questo Governo ha dimostrato grandissima sensibilità verso questi temi. Il nostro Ministro dell'interno è più volte intervenuto e ha assicurato che ci sarà un'azione del Governo in questa direzione.

oggi stiamo dando. *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui riuniti oggi per affrontare la discussione di un importante disegno di legge, che nasce dallo straordinario lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, presieduta dalla senatrice Lo Moro, prima firmataria del disegno di legge, che saluto e ringrazio calorosamente. Se c'è un tema che mi sta particolarmente a cuore e per il quale sento l'obbligo di battermi, questo è proprio quello della tutela degli amministratori locali che ogni giorno, stoicamente, compiono il loro dovere civico negli oltre 8.000 Comuni italiani. Dal rapporto della Commissione sono purtroppo emersi numeri sconfortanti, che hanno restituito la fotografia di un Paese nel quale i rappresentanti delle istituzioni sono costantemente minacciati. Ogni giorno infatti vengono registrati quasi tre episodi di violenza o di intimidazione. Centotrentadue omicidi negli ultimi quarant'anni, dieci solo nell'ultimo decennio, sono i numeri di una guerra lunga e silenziosa

Giuseppe Valarioti, Marcello Torre, Domenico de Maio, Angelo Vassallo, Pasquale Grillo e tanti altri sono state vittime di questa guerra. I loro nomi sono finiti sulle cronache di giornale e ancora oggi, dopo decenni, li ricordiamo come martiri civili del nostro Paese. Ma sono migliaia le storie di minacce e intimidazioni che non si concludono tragicamente e, pertanto, rimangono sconosciute, senza arrivare all'attenzione dell'opinione pubblica, sia perché manca il coraggio di denunciare, sia perché gli strumenti legislativi sono stati, finora, troppo deboli Gli amministratori locali sono l'avamposto delle istituzioni sul territorio, la cartina di tornasole di un rapporto tra cittadini e Stato non sempre facile, né del tutto trasparente. Nei loro confronti si verificano minacce e aggressioni sia di carattere punitivo che preventivo, solo così si spiega perché vengono colpiti sia ex amministratori, puniti per ciò che hanno o non hanno fatto, sia politici e candidati, avvertiti preventivamente sulle conseguenze delle loro azioni. E se è vero che buona parte delle violenze sono legate alla criminalità organizzata, dietro tante intimidazioni c'è anche altro: interessi economici, malaffare, fenomeni corruttivi sempre tristemente alla ribalta della cronaca e agli interessi personali di varia natura che si muovono nella

Sapeva bene che l'utilità ricavata nel rapporto con il politico corrotto si traduce in appalti dirottati, abusi sui permessi edilizi, posti di lavoro non dichiarati e tutelati, concessioni che interferiscono sistematicamente sull'attività amministrativa pubblica, che, in forza dello scambio politico mafioso, viene orientata a soddisfare gli interessi di pochi (gli amici degli amici) piuttosto che al perseguimento dell'interesse generale e pubblico. Di tutto questo ne abbiamo prove talmente evidenti, anzitutto a livello ambientale. È il caso del dissesto idrogeologico con l'usura del suolo, frane, smottamenti e allagamenti dovuti all'abbandono del territorio e alla mancata cura dei versanti; della cementificazione selvaggia senza regole, con case non costruite secondo norme antisismiche e con materiali scadenti tanto da sbriciolarsi alla prima scossa di terremoto; delle infrastrutture statali poste su pendii talmente instabili da franare al passaggio dei treni; degli interi Paesi sviluppatisi in alvei di fiumi che, con le piogge abbondanti, vedono correre nelle loro strade metri cubi di acqua determinando perdite di vite umane. Finalmente, quindi, il Parlamento ha deciso,

Per questo motivo plaudo alle modifiche proposte dal disegno di legge, che consentiranno una più penetrante ed efficace azione giudiziaria, un utilizzo di tutti i più importanti strumenti di indagine, delle aggravanti generiche e dell'arresto in flagranza di reato per coloro i quali si macchieranno di reati di intimidazione o ritorsione, sia nei confronti di amministratori locali che di candidati a cariche elettive. Mi auguro, quindi, che questo sia un primo passo affinché lo Stato possa garantire una maggiore presenza, anche fisica, delle istituzioni nazionali al fianco degli amministratori locali. Il passo futuro dovrà essere quello di rafforzare programmi di prevenzione e di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, i cui organici, come ben come ben sappiamo, non sono adeguati alle esigenze. Sarà poi necessario istituire una banca dati nazionale per la rilevazione degli episodi intimidatori e il loro censimento, alimentata e condivisa dai diversi soggetti impegnati nella repressione di tali reati. Oggetto di accertamento dovrebbero essere anche le dimissioni, individuali o collettive, di amministratori comunali, specie quando esse diano origine allo scioglimento di un Consiglio comunale, soprattutto se si considera che una quota rilevante delle dimissioni dalla carica Si dovrà poi realizzare un maggior coordinamento tra amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la magistratura e gli enti territoriali, che permettano all'amministratore locale di avvalersi dell'apporto di altre competenze in un quadro di assoluta trasparenza e ricostituire e ricostituire un clima di fiducia nelle istituzioni rappresentative. Le rilevanti responsabilità che finiscono per ricadere sul sindaco - nella gestione del territorio, nelle gare di appalto, nella concessione delle licenze e dei sussidi, nel ciclo dei rifiuti o nella gestione dei beni confiscati rendono necessaria una semplificazione della normativa al fine di chiarire, anche di fronte all'opinione pubblica, quali siano le competenze dei rappresentanti politici e quelle dell'apparato amministrativo e rendere più snelle le procedure. In materia di appalti, occorrerebbe attribuire le responsabilità gestionali amministrative ad altri livelli istituzionali, collocati più in alto, soprattutto per sgravare i Comuni più piccoli, che si trovano troppo spesso in difficoltà nei confronti di poteri molto forti. Vorrei accennare, con estremo rammarico, a un altro tema, anch'esso

politici e funzionari pubblici, che produce violenza e sfiducia. Un'autentica minaccia per la democrazia che possiamo sconfiggere solo comportandoci in in maniera retta e trasparente. D'altro canto, cari colleghi senatori, solo impegnandoci seriamente per presentare ai cittadini liste e candidature integerrime, lontane da qualsiasi legame con la criminalità organizzata e il malaffare, potremo recuperare quella crisi di fiducia che ha investito la classe politica italiana. In un quadro generale di sfiducia nella politica, chiunque sia stato anche solo sfiorato da vicende che lo possano avvicinare alle mafie dovrebbe fare un passo indietro per il bene di tutti. Concludo dicendo che ho voluto ricordare i nomi di alcuni amministratori locali uccisi perché fortunatamente ci rammentano che non c'è solo una politica che spesso viene descritta come collusa e connivente, ma che ci sono stati e ci sono donne e uomini che sanno interpretare, fino alle estreme conseguenze, il senso vero dell'impegno politico e civile. Le intimidazioni sono contro gli amministratori per bene, quelli che non si piegano a nessun volere, e solo in minima parte entra nel mirino chi non ha rispettato gli accordi. questo per dire che non tutta la politica è uguale. Mi auguro che con il disegno di legge in esame si possa offrire una maggiore tutela agli amministratori di tutta Italia, affinché possano compiere il loro lavoro serenamente, onestamente e a favore di tutti i cittadini.

il disegno di legge di cui si sta discutendo oggi in Assemblea ha un'importanza storica se solo si considerano le grandi battaglie, condotte ormai da decenni, contro le mafie e per lo sviluppo della nostra comunità.

Sappiamo benissimo che, come del resto emerso anche nel corso delle audizioni condotte durante l'attività della Commissione, sempre più spesso tanti che hanno scelto di candidarsi o di amministrare i diversi Comuni su cui si fonda la nostra Repubblica avvertono un sentimento di solitudine o di distanza dallo Stato nel libero esercizio del potere di rappresentanza o di governo di un'autonomia locale. perché le forme e le connotazioni delle pressioni o delle intimidazioni possono essere le più varie e oscure. Questo sentimento, che non sempre è accompagnato da atti eclatanti, produce disimpegno, sfiducia e rassegnazione non solo in chi amministra, ma, in generale, nel tessuto più profondo delle nostre comunità,

sono costretti a subire aggressioni o violenze solamente perché non vogliono assecondare gli interessi particolari, spesso illeciti, o perché provano a contrastare la penetrazione della criminalità nelle istituzioni, dando prova di buon governo e di forte etica del dovere. La storia del nostro Paese - non solo del Mezzogiorno, purtroppo ci racconta anche di vite distrutte, auto incendiate e famiglie colpite perché le mafie provano sempre a sfidare lo Stato. Il Rapporto 2014 «Amministratori sotto tiro», pubblicato dall'associazione

tra minacce dirette e indirette, spesso con sostanziale impunità e ripetitività degli atti di violenza; seguono il Nord con il 14 per cento e il Centro con il 12 per cento dei casi. Non possiamo in alcun modo permetterci alcuna sottovalutazione del fenomeno, né sul piano della ricerca dei moventi, né su quello di un più adeguato intervento normativo. Solo pochi giorni fa, in occasione del settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, il presidente Mattarella ha espresso un forte richiamo all'assoluta priorità di un contrasto incisivo alle mafie, evidenziando come «l'efficacia e la credibilità dell'azione pubblica si fondano sul rispetto della legalità, sull'etica del servizio e sulla trasparenza» e che «occorre grande fermezza contro ogni tentativo di asservire uffici e istituzioni a interessi personali, favoritismi e malaffare». Fare politica trasparente in molte delle nostre realtà è certamente rischioso, perché richiede passione civile e responsabilità individuale. E c'è un ulteriore aspetto che merita di essere approfondito: troppo spesso la piaga della "intermediazione impropria" dei politici, la tentazione di trasformare i diritti dei cittadini in favori concessi solo ad alcuni e negati ad altri, ai fini esclusivi del consenso, è alimentata da una cattiva politica, che molto spesso entra in contatto con le organizzazioni criminali, creando intrecci perversi in cambio di assunzioni, di gare d'appalto pilotate, di licenze, sovvenzioni o contributi agevolati. In questo quadro, la crisi economica, che alimenta ansie e incertezze, condiziona paure e bisogni, rende le autonomie locali, già gravate da difficoltà finanziarie e risorse disponibili sempre più scarse, il primo interlocutore del cittadino in cerca di protezione e sostegno. Per spezzare questo circuito, parallelamente alle puntuali modifiche delle norme penali ipotizzate dal disegno di legge in esame, occorre continuare in un ottica sistemica, da un lato, a lavorare per promuovere una buona politica orientata all'interesse generale e, dall'altro, a migliorare la qualità della pubblica amministrazione, dando nuova centralità alla trasparenza La grande novità del disegno di legge che stiamo esaminando, però, sta proprio nel tentativo coraggioso di creare una fortissima barriera, che impedisca ogni tipo di contatto o rapporto tra gruppi di pressione criminale e gli amministratori locali, dando una visione finalmente unitaria al fenomeno intimidatorio, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione. Ad oggi infatti, specialmente nei settori di maggiore vulnerabilità, oggetto di potenziale interesse delle mafie, la normativa esistente ha mostrato tutti i suoi limiti, pur in presenza di concreti indicatori di pericolo, che pregiudicano la libera determinazione della democrazia rappresentativa. In conclusione, la grande sfida di cambiamento radicale che una politica riformatrice deve saper realizzare è esattamente questa: liberare le potenzialità della società e dell'economia contrastando con efficacia

Del resto, la qualità della nostra democrazia sarà migliore se riusciremo davvero a tutelare quei consiglieri comunali o quegli amministratori che provano con onestà ad esercitare il mandato ricevuto dai propri cittadini attraverso il voto democratico.

per approvare il disegno di legge in esame, che introduce modifiche normative in materia penale. In particolare viene modificato l'articolo 338 del codice penale, che prevede il reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, in modo da adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela degli amministratori locali. Tale fenomeno costituisce una realtà gravissima, un *vulnus* all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa. Convivere con il timore di rimetterci la pelle da parte dei pubblici funzionari, nell'esercizio dei propri doveri e delle proprie funzioni, genera danni alla tenuta complessiva del sistema Paese.

e si trovano spesso nella condizione di subire gravi atti di prevaricazione e strisciante ricatto tanto che i loro familiari temono per la propria incolumità. Tutto ciò si traduce in insicurezza sociale, territori segnati da illegalità, fuga di capitali e di intelligenze, allontanamento degli investitori dalle comunità destinatarie di providenze, instabilità amministrativa, mortificazione della politica quale campo di esercizio

ritardo di sviluppo e drastica diminuzione di prodotto interno lordo. Innumerevoli sono ogni anno gli atti di sindacato ispettivo presso Camera e Senato con cui si sottolineano tali situazioni e si richiedono misure di protezione. Questo intervento legislativo sicuramente costituisce un passo nella direzione di una disciplina più rigida e determinata al contrasto

prevedere delle aggravanti e degli aumenti di pena non siano, da sole, misure sufficienti, nella pratica, a contrastare efficacemente, ma soprattutto a prevenire la commissione dei reati penali, se non sono accompagnate dalla certezza della pena, cioè dalla certezza della erogazione della sanzione penale. penale. Infatti il fondamento di un ordinamento giuridico moderno, è costituito, non dal fine coercitivo delle norme, ma prima ancora dal loro carattere preventivo, cioè dalla "certezza del diritto" che imprescindibilmente si declina nella "certezza della pena" che è il vero deterrente. Perciò non è superfluo ricordare che è questa la malattia terminale del nostro Paese. Questa è la causa dell'inefficacia del nostro sistema penale e di ciò occorre prendere coscienza. Non basta scrivere le leggi, anche se sono delle buone leggi, se poi chi delinque sa che comunque resterà impunito e sarà vano il tentativo dello Stato di ristabilire legalità, legittimità, cura della libertà, dei diritti e dei doveri.

Signora Presidente, la prima questione che dobbiamo tutti porci è se sia necessario o meno intervenire in questa materia per il contrasto ad azioni criminali nei confronti di amministratori locali. Io credo di sì, sono fermamente convinto della necessità di un intervento legislativo. Non condivido invece la tecnica utilizzata per pervenire al risultato. È notorio che l'articolo 338 del codice penale prevede la configurazione di un reato quando vi è un'azione di violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Da una giurisprudenza risalente al 1954 e ribadita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. sentenza n. 5611 del 2012, anche l'ipotesi di una minaccia ad un componente del corpo politico, amministrativo o giudiziario è fattispecie ritenuta compresa nell'articolo 338. In particolare,

cui dirò dopo e di cui parlava il relatore - e, nella specie, la deliberazione di costituzione dell'ente comunale quale parte civile nel processo nei confronti dell'imputato.

nel tempo il chiarimento giurisprudenziale secondo cui, per la sussistenza del reato in esame, non è necessario che la minaccia sia fatta in presenza dell'organo collegiale riunito, essendo invece sufficiente la cosciente volontà da parte dell'agente di dirigere la minaccia ad un corpo con lo scopo di impedirne o turbarne l'attività, cosicché anche la minaccia rivolta ad uno dei suoi membri assume decisiva rilevanza. La Corte richiama in proposito una sentenza del 1954. Non nego che vi sia un'altra giurisprudenza della Corte di cassazione, che non ho mai condiviso, che non ritiene possibile la configurazione nei confronti che fa riferimento anche ai singoli componenti, andiamo a riconoscere fondamento a quella giurisprudenza che negava la possibilità di configurare, con una possibilità di intervento anche sui procedimenti in corso. E questa è una cosa che io non voglio. Pertanto, ho utilizzato l'articolo 336 del codice penale per inserire la stessa identica norma prevista dal testo del disegno di legge. Non è una questione politica, ma una questione solo tecnica

finalizzati a: «ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Per tali

come nell'esempio, cui ho fatto riferimento, della sentenza della Corte di cassazione. Quella condotta è già prevista e non può essere una condotta del codice penale: il reato di diffamazione. Ma se il connotato è la violenza o la minaccia, allora in quel caso è previsto comunque.

che rafforzi il contrasto verso chi agisce nei confronti degli amministratori locali o, per una questione di principio e non di tecnica né di politica,

È questo ciò che mi preoccupa di più: legittimare una interpretazione che avevamo tentato di contrastare. Mi domando perché non sia possibile

Noi siamo per l'approvazione di una norma che abbia un'effettiva efficacia di deterrenza, che non crei problemi interpretativi da parte della giurisprudenza e, nello stesso tempo, garantisca una punizione effettiva una punizione effettiva di determinati comportamenti. Per cui, anche sotto il profilo della pena, non muta la valutazione ai

Non potete pensare di fare un'aggravante che costituisce la stessa condotta, quindi prevedendo una duplice possibilità di condanna. Per questa ragione, signor Presidente, confido

onorevoli senatrici, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, come è stato ben sottolineato dal relatore, senatore Cucca, il disegno di legge trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, di cui sono stata onorata onorata di essere componente, che ha concluso la propria attività nel febbraio 2015 e ha prodotto il disegno di legge di cui sono cofirmataria. Guidati dalla presidente, senatrice Doris Lo Moro, abbiamo verificato in quale misura fosse congrua la normativa vigente rispetto alle problematiche analizzate abbiamo proposto soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto al fenomeno, così da assicurare il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. Ricordo che la Commissione ha attivato la propria indagine sull'intero territorio nazionale e, pur con diverse matrici e dinamiche che connotano le aree geografiche, si è convenuta, nelle indicazioni finali, la necessità di affrontare il tema con una visione unitaria, cogliendo gli elementi comuni che lo caratterizzano e, in particolare, approfondendo la qualità soggettiva della vittima e indagando sulla finalità dell'azione intimidatoria. Oggi diamo una prima importante risposta, un atto doveroso nei confronti di tutti quegli amministratori e funzionari pubblici che quotidianamente vengono messi sotto pressione o minacciati per condizionarne l'attività amministrativa. Abbiamo ascoltato le loro testimonianze e individuato campi di azione e strumenti di sostegno. Scegliamo, per questo, come primo intervento, di inasprire le pene. Diamo un segnale forte a chi cerca di contrastare senza scrupoli l'operato di coloro che lavorano correttamente a difesa e nell'interesse della collettività. Diciamo agli amministratori locali esposti in prima persona che non sono soli. Si tratta di un impegno che deve riguardare tutti i tipi di pressione illecita, non solo quelle di stampo mafioso, riferendoci a tutti gli organi amministrativi, esecutivi e di indirizzo, per gli esponenti di maggioranza come pure di minoranza, per i dirigenti e i funzionari

I sindaci ci chiedono di essere al loro fianco anche nei difficili *iter* autorizzativi. La presenza dello Stato e dei diversi livelli di governo (regionale, provinciale) sono determinanti per dar forza alle scelte politiche a tutela dei territori e di talune aree di pregio (penso alle aree protette del Ticino, del lago Maggiore e delle Lame del Sesia). Le stesse amministrazioni si stanno attrezzando, cogliendo appieno la necessità di strutturare difese forti. La Provincia di Novara, unica in Piemonte, si è dotata di un piano cave che definisce quantità di materiale estraibile e bacini di estrazione; la prefettura si è attivata, anche a seguito dei gravi episodi verificatesi in anni recenti, con un protocollo di legalità per il controllo e il monitoraggio delle cave sottoscritto dal prefetto, dal procuratore della Repubblica, dalla Provincia, da decine di Comuni, dall'ARPA, dalle Forze dell'ordine, dalla direzione territoriale del lavoro, dall'ASL e dalle rappresentanze delle categorie degli operatori nel settore delle attività estrattive e del trattamento dei rifiuti. La Regione Piemonte, proprio in questi mesi, sta lavorando ad una nuova legge, promossa dal Gruppo del Partito Democratico a palazzo Lascaris, sulle attività estrattive: una norma che si fa carico anche del sostegno agli amministratori, a partire dalla programmazione a livello regionale delle attività estrattive, per superare le disuguaglianze territoriali che penalizzano

e dei rifiuti è un settore che trova corrispettivi di fragilità anche in altri ambiti del sistema amministrativo, come quello della gestione dei servizi socio-assistenziali, delle politiche abitative, dei trattamenti sanitari obbligatori, degli interventi di abbattimento di edifici abusivi, attività svolte in pieno rispetto della legge e della trasparenza, ma che necessitano di una rete di protezione nei confronti dei sindaci e dell'apparato. Durante i lavori della Commissione abbiamo raccolto una spinta dal basso, che ci chiede di continuare sulla strada della tutela degli amministratori pubblici, con normative volte a intervenire su aspetti organizzativi e amministrativi, prevenendo la solitudine Non abbassiamo la guardia e mettiamo in campo convintamente e con senso di responsabilità ogni strumento utile per consentire agli amministratori di proseguire con maggiore serenità la loro fondamentale attività di governo dei territori. Il disegno di legge in esame si riferisce - come si diceva - alle ipotesi di modifiche normative in materia penale emerse nella Commissione di inchiesta, con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione dell'evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione dell'integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato). La modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, è quindi individuata ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela. Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte. Tutto ciò consentirà di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, e in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno a sette anni) che consente il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e ad ogni altro mezzo di prova. La Commissione ha inoltre suggerito una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è possibile procedere all'arresto in flagranza di reato. In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, cioè a quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, si è ravvisata l'esigenza di prevedere una nuova circostanza ad effetto speciale, che prevede un aumento di pena qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Da qui è evidente quanto il disegno di legge in discussione impatti con la reale vita democratica del Paese e di fatto costituisca un importante rafforzamento della tutela degli amministratori locali dei funzionari appartenenti al corpo amministrativo e giudiziario. Vorrei chiudere il mio intervento con il ricordo di Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo, assassinata nel suo ufficio, in Comune, da un vigile sospeso dall'incarico. Per la prima volta il Comune lombardo aveva eletto una donna come prima cittadina. E proprio in questo contesto, ancora grondante di sgomento e dolore, abbiamo onorato la sua memoria, svolgendo un'audizione della Commissione d'inchiesta. Dedico a lei questo mio intervento a sostegno dell'approvazione del disegno di legge in discussione. Signor Presidente, dobbiamo ringraziare la Commissione d'inchiesta, la sua Presidente e tutti i componenti

Colleghi, non stiamo qui trattando una fattispecie penale che lascia il tempo che trova, o non stiamo facendo un esercizio retorico a favore del corpo politico dello Stato: qui stiamo dando una risposta vera e reale a una minaccia, a una violenza ripetuta e sistematica che si abbatte sui nostri amministratori, quotidianamente, giorno per giorno, in tutti i territori. Cari colleghi, immaginate se in un altro Paese a democrazia avanzata avvenisse lo stesso fenomeno; ci sarebbe una mobilitazione. La democrazia saprebbe trovare il rigore per bloccare il tentativo di di deviare, di condizionare e umiliare la democrazia locale. Ecco perché l'unico rimprovero che si può fare al Parlamento è che siamo arrivati in ritardo.

Ecco l'intervento che è stato fatto: un intervento di chirurgia cui è sottesa la capacità di attivare una norma penale che deve finalmente svolgere la sua funzione di deterrenza, per impedire, anche nel 2016, che tanti amministratori esposti subiscano minacce e violenze. Attenzione, cari colleghi, parliamo anche di casi in cui sono state rovinate delle persone o rese invalide; molti hanno anche perso la vita. Stiamo parlando quindi non solo delle classiche minacce, come il foglietto che arriva,

a quella condivisione che è stata raggiunta nella Commissione d'inchiesta e alla comune valutazione che è stata raggiunta in Commissione giustizia per proporre lo spostamento della condotta da punire all'articolo 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che già oggi

inoltre nelle condizioni d'intervenire con intelligenza sulle circostanze aggravanti, naturalmente senza creare contraddizioni. tuttavia, è comparsa una contraddizione: ci è stato spiegato che potremmo ledere il diritto dei cittadini a essere informati, quindi anche intervenire contro la libertà d'informazione.

c'è assolutamente. Tuttavia, per fugare qualunque dubbio ed evitare che attorno a questo tema molto sensibile e caro a tutti noi si possa scatenare, come spesso avviene nel nostro Paese, una serie di interpretazioni forzate e un po' maliziose che si macchiano poi anche di un certo spregevole interesse e conflitto politico (che in questi casi non ha ragione di essere), il relatore ci ha proposto un'ulteriore riformulazione che ci mette nelle condizioni di allontanare

per migliorare ulteriormente il testo e fare in modo che ci si allontani ancora di più da qualunque interpretazione nel senso di mettere in discussione il diritto all'informazione. Apprezziamo quest'apertura da parte del relatore. Il Partito Democratico è pronto a dare il suo contributo; lo vuole fare insieme a tutti gli altri Gruppi, al Presidente della Commissione giustizia, alla Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno

da condividere tutti e da presentare positivamente al Paese, per fare in modo che la democrazia locale dispieghi tutte le sue energie, senza interferenze causate da azioni di minaccia o di violenza tali da colpire singole personalità che fanno parte del corpo politico, amministrativo e giudiziario del nostro Paese e fare in modo così che la democrazia, che si articola nei differenti poteri, possa trovare quella fisiologica energia e forza che in un Paese come il nostro diventa anche vitalità democratica. Signor Presidente, siamo quindi pronti a passare successivamente alla fase emendativa a fare in modo che tutti i contributi siano valorizzati. Ringrazio il Governo che ha dato la sua disponibilità, ci ha accompagnato ed è pronto a dare anche il suo apporto. Alla fine avremo un testo fatto bene, sistematico e in grado di dire al Paese: giù le mani dalla democrazia, giù le mani dalla vita della democrazia. La democrazia si svolga nella sua fisiologia, abbia i suoi momenti di contrapposizione, ma mai la violenza e la minaccia possono essere uno strumento di regolazione del rapporto tra i territori e la vita democratica del nostro Paese. Ecco perché siamo pronti a dare il nostro contributo e siamo convinti che alla fine troveremo la giusta convergenza e tireremo fuori un ottimo testo.

il tema delle intimidazioni agli amministratori locali è particolarmente sentito dal sottoscritto oltre che dall'intero Gruppo che oggi ho l'onore di rappresentare in Senato, i Conservatori e Riformisti. Da anni, ormai, fare il sindaco, l'assessore o il consigliere comunale è diventata una vera e propria missione e una difficile sfida, se pensiamo che alle normali problematiche da risolvere si sono aggiunti tagli e ristrettezze finanziarie. Troppo spesso, come dicevo, in nome e per conto di quella missione civica, essi subiscono intimidazioni fuori dalla norma. Che si tratti di parole o peggio ancora di gesti, il senso di questi gravi atti non cambia perché il fenomeno non può essere né ammesso né mai sottovalutato. È necessario pertanto che le istituzioni, a tutti i livelli, non si limitino a mere dichiarazioni di vicinanza e solidarietà, ma sostengano concretamente gli amministratori che svolgono il proprio compito per la legalità e per le proprie comunità. Per tali ragioni e per quanto accennato, avverto la necessità di farmi portavoce di un'esigenza che non tocca solo la sicurezza delle cariche pubbliche, ma anche il senso stesso di civiltà e modernità della della democrazia negli enti locali italiani. Mi auguro pertanto che questa Camera sappia qui fornire una risposta tangibile e un sostegno finalmente concreto e attuabile ai tanti amministratori locali, che da Nord a Sud lo chiedono a gran voce. Voglio in questa sede ricordare che nel 2013 è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Tale Commissione ha avuto il pregio di monitorare e quantificare il fenomeno tra il 1° giugno 2013 e il 30 aprile 2014. Il lavoro è stato poi proseguito dall'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dell'interno il 2 luglio 2015. Quanto è emerso, colleghi, è allarmante. Gli atti di intimidazione, rilevati sull'intero territorio nazionale, sono stati 668 nel 2013 805 nel 2014. Nel 2015 c'è stato un lieve calo (619), ma la sostanza e la gravità della situazione è stata in pratica la stessa. Ciò di cui parliamo è ancor più complesso se pensiamo che spessissimo le sue cause non sono riconducibili a presunte colpe della politica locale (mancanza di lavoro *in primis*). Su questo fronte, purtroppo la mia Regione, la Puglia, è una delle più colpite, seconda solo alla Sicilia.

assessore del Comune di Nardò, in provincia di Lecce; di Gianni Carnicella nel 1992, sindaco di Molfetta, in provincia di Bari;

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, è pertanto di enorme rilevanza per il bene delle nostre comunità. Il suo testo fortunatamente modifica l'articolo 338 del codice penale, colmando così un vuoto di tutela che si era fino ad oggi protratto avendo causato danni a tanti onesti cittadini e loro famiglie. Non dimentichiamo infatti che dietro le minacce ad un amministratore c'è sempre anche il dolore di figli, mogli, mariti e parenti, ancora più incolpevoli. Ma tornando al testo, è possibile dire, concludendo, che costituisce una prima risposta. È però necessario fare e pretendere di più, su tanti livelli. Penso per esempio a modalità serie per l'uso della videosorveglianza al fine di prevenire la commissione di questi gravissimi reati soprattutto nei piccoli centri, periferici e dimenticati. *Idem* dicasi sullo snellimento delle tante procedure burocratiche tortuose che lasciano spesso soli sindaci e assessori di fronte ad immotivati atti di prepotenza. Non dimentichiamo neanche, anche se non sono tecnicamente amministratori, i tanti dirigenti, funzionari e impiegati che svolgono in silenzio il proprio lavoro e che risultano a volte parte Il tema meriterebbe molto più tempo e spazio, ma ora passiamo dalle parole ai fatti. Comprendiamo noi stessi in questa sede che *in primis* non è più possibile considerare tale fenomeno come una questione di serie B e che ad esso è legato la crescita «normale e serena» delle nostre comunità locali. Impegniamoci perché da questi atti passi anche un doveroso messaggio alle nuove generazioni verso il sano impegno per la politica, che è e deve sempre continuare ad essere passione e dedizione libera e incondizionata nei confronti dei cittadini. Per quanto sopra esposto, apprezziamo lo spirito del testo, seppur ribadendo che si deve trattare solo di un primo passaggio verso la definitiva presa d'atto e soluzione del problema. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

eppure, siamo arrivati fino ad oggi con delle norme che probabilmente non sono state sufficienti a combattere il fenomeno delle intimidazioni verso organi politici e, in particolare, amministrativi.

per arrivare a una proposta normativa che, per alcune parti, condividiamo. Sono preoccupanti i dati relativi ai fenomeni di intimidazione verso, in particolare, gli organi amministrativi.

dal recapito di proiettili, parti di animali, ordigni o lettere minatorie, a incendi di autovetture o altri beni di proprietà degli amministratori.

quasi di favore nei confronti di un organo politico nel momento in cui vengono perpetrati dei reati a suo danno. Riteniamo - ovviamente

Signor Presidente, ho cercato di seguire con attenzione il dibattito, ma per l'ennesima volta devo dire che, sentendo i colleghi parlare, mi sono domandato di cosa stessero parlando. c'è un fenomeno allarmante, su cui bisogna intervenire, che è quello delle aggressioni e delle minacce agli amministratori locali. Del resto, anche in Commissione il provvedimento che stiamo discutendo era intitolato: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali».

Ricordo, nel periodo 1992-1994, le difese che feci quando c'era la criminalizzazione generalizzata degli amministratori locali, rispetto a situazioni che ho vissuto di persona. Sono andato a trovare le vedove di amministratori e sindaci che hanno perso la vita perché qualche amministrato li aveva colpiti e uccisi, non avendo avuto da loro quello che si aspettava di avere. Quindi, quando ho sentito i colleghi parlare della necessità di intervenire per tutelare gli amministratori locali, ho detto che ero perfettamente d'accordo. Se il testo che stiamo discutendo fosse quello, lo voterei: peccato che il testo sia tutt'altro. testo che stiamo discutendo e che voteremo non riguarda soltanto gli amministratori locali, ma riguarda «anche» gli amministratori locali. Non capisco perché nessuno tra i colleghi del PD abbia fatto riferimento al fatto che, addirittura, il titolo del provvedimento sia stato modificato all'ultimo secondo, perché agli amministratori locali si sono aggiunti i singoli componenti dei corpi politici, amministrativi e giudiziari

accorti di questo tentativo. Ricordo ai colleghi che i parlamentari, per fortuna, nella Costituzione hanno una garanzia: non sono chiamati a rispondere delle opinioni espresse. Tutti sappiamo che se un cittadino ci querela o ci intenta una causa civile per le cose dette in Assemblea, in Commissione, o anche fuori se queste hanno un collegamento con l'attività parlamentare, l'azione di questo cittadino viene paralizzata, perché il parlamentare ha una tutela giudiziaria, che naturalmente il cittadino non ha, nei confronti del parlamentare, che lo può viceversa querelare e gli può intentare causa civile. I magistrati hanno una "piccola" particolarità rispetto al cittadino, al giornalista comune o anche la parlamentare: chi decide sulle cause di diffamazione o sulle cause civili che riguardano i magistrati, sono Basta andare a vedere i tempi delle querele e delle cause civili che riguardano i magistrati e quello che ricavano da queste cause, per accorgersi che, inevitabilmente, il fatto che siano i magistrati a decidere su questioni che riguardano i magistrati - i dati sono lì

una loro opinione, che noi riteniamo diffamatoria, nei confronti dell'attività del Parlamento, di un legislatore o dell'attività di un magistrato.

passiamo a situazioni di fatto che vanno colpite. Ma nel momento in cui parliamo semplicemente di minacce o di o di atteggiamenti che riteniamo diffamatori nei confronti di magistrati o di parlamentari andiamo su un piano assolutamente diverso, come andiamo su un piano diverso quando all'articolo 1 aggiungiamo

e noi voteremo «no» al *referendum*: è una ritorsione. È una minaccia ritorsiva. Rientra in questa legge, visto che un emendamento del relatore prevede

o oggetto di azioni ritorsive possa fare come qualsiasi altro cittadino, e cioè ricorrere alla magistratura per tutelare i suoi diritti. Qualcuno mi deve spiegare - e nessuno l'ha fatto perché tutti i colleghi che hanno parlato finora hanno parlato di amministratori locali - perché queste norme si estendono anche ai parlamentari e ai magistrati e perché i parlamentari e i magistrati devono essere più uguali degli altri cittadini. Come si fa a qualificare una campagna di stampa o degli articoli come ritorsivi?

noi, come principio teorico, aggraviamo le pene per chi ha questo tipo di atteggiamento nei confronti dei parlamentari e dei magistrati, lasciando così i cittadini in secondo piano.

Si elimina il riferimento ai parlamentari e ai magistrati e la si vota per tutelare gli amministratori locali dalla diffamazione, dai danneggiamenti, dalle minacce e da tutto ciò che li mette in difficoltà sul territorio.

dopo che i loro congiunti, che svolgevano un'attività pubblica così onerosa e difficile come quella di chi si confronta con il territorio, hanno pagato il loro servizio alla comunità. Non vorrei però confondere le due sulla base di quanto accadrà domani e dell'accoglienza che riceveranno i nostri emendamenti, noi parametreremo il nostro voto finale su questo

un lavoro importante. La Commissione d'inchiesta sugli attentati e sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali è stata voluta da subito.

e sociale, e che, anche in ragione di fenomeni di ribellismo disordinato, e non solo in relazione a vicende di criminalità organizzata, oggetto di intimidazioni e di attentati, insieme alle loro famiglie. Il lavoro svolto dalla Commissione è stato importante, perché questo tema è stato sviscerato in tutti i suoi diversi aspetti

Ci sono situazioni nelle quali le amministrazioni locali sono interpretate come una presenza oppressiva dello Stato. Ci sono altre situazioni nelle quali le amministrazioni locali sono considerate complici di attività criminali e sono oppressive nei confronti dei diritti della cittadinanza. Ci sono situazioni nelle quali comunità sane sono aggredite dall'esterno da fenomeni criminali che si sono insediati a seguito di interventi destinati a coltivare interessi, in genere sempre molto precisi, di natura economica,

illiceità e sono espressione di comportamenti disonesti. quindi, non è un disegno di legge che tende a difendere il personale politico qualunque esso sia. È piuttosto un disegno di legge che intende affermare l'autorità dello Stato anche nelle sue articolazioni locali. Ed è proprio attraverso l'affermazione dell'autorità dello Stato e della società organizzata, secondo i principi della Costituzione, in funzione della civile convivenza, della ricerca del benessere comune e della difesa del bene comune,

da chi lo attacca con le intimidazioni violente e con gli attentati alle cose, anche pubbliche, anche del Comune, anche di proprietà dello Stato, dello Stato, per condizionarne i comportamenti, per renderne difficile la funzione, per incutere paura, timore

- approvato, anche con le modifiche che riteniamo siano più giuste per sgombrare il campo dall'idea che sia che sia un provvedimento difensivo del corpo politico corrotto, decomposto.

chi fa politica abbia qualcosa che non va. Se c'è una mela bacata dentro il cesto, quella si orienta a fare l'amministratore locale, a candidarsi al Parlamento o al Governo del Paese.

partendo da esempi certamente negativi, che noi possiamo riscontrare nella politica come nelle professioni, come nell'economia, come nella vita quotidiana della nostra società, in tanti rami dell'attività umana. E penso anche che chi esercita la funzione politica abbia più responsabilità. Ma non esiste una società civile, se non c'è una società organizzata, se non esiste uno Stato, se non esiste un'autorità democraticamente individuata, che esercita le funzioni pubbliche di tutela e garanzia delle libertà di ciascuno di noi. Non esiste. Esiste un'anarchia dei più forti. E chi ha in mente di colpire la funzione politica, anche attraverso le intimidazioni che si esercitano nei confronti dei nostri amministratori locali (quelli che vivono la condizione più periferica),

È questo che noi dobbiamo difendere, anche attraverso questo provvedimento. Mi si dice che l'articolo 3 è discusso e anche discutibile, perché individuerebbe nell'articolo 595 del codice penale una regolazione diversa delle pene in funzione della della diffamazione mirata a colpire l'amministratore locale o piuttosto il funzionario pubblico, anche quello impegnato nel ramo della giustizia.

è uno dei temi che si è trattato, che si è voluto trattare e che si è ampiamente discusso, per esempio

È un'invenzione che viene direttamente dagli operatori dell'informazione, da autorevolissimi esponenti del settore della comunicazione. Quindi, quando si dice che la macchina del fango è usata e può essere usata in modo funzionale per colpire gli operatori pubblici, gli amministratori locali, i funzionari onesti e gli amministratori della giustizia, noi dobbiamo difenderli e in qualche modo bisogna che li difendiamo. Se pensiamo che la diffamazione, cioè la macchina del fango, sia un nemico, lo dicano prima di ogni altro coloro che hanno indicato la macchina del fango come uno degli strumenti più utilizzati per colpire l'azione onesta dei nostri amministratori onesti e operatori pubblici. Noi dobbiamo uscire dall'emergenza nella quale abbiamo vissuto negli ultimi anni, e dobbiamo trovare il modo. È giusto che teniamo gli occhi bene aperti per trovare ciò che di illecito si fa all'interno dei rami dell'amministrazione pubblica, nel funzionamento dello Stato, perché esso deve garantire i cittadini e come tale non può essere inquinato. Al contempo, però, dobbiamo avere la responsabilità di difendere sempre di più e restituire, in quest'azione di difesa, il prestigio che meritano coloro che si impegnano per tutti e lo fanno attraverso la loro azione nelle istituzioni democratiche, nel sistema delle autonomie, negli uffici pubblici e nell'organizzazione e amministrazione della giustizia. Dobbiamo avere il coraggio. Non dobbiamo più accedere all'idea che tutti siamo uguali, perché non è vero. È una falsità. E coloro che indicano, in modo qualunquista, lo fanno per interesse, e non perché si sbagliano; lo fanno perché l'hanno pensato, l'hanno organizzato lo gestiscono in quella funzione: smantellare lo Stato democratico è l'obiettivo di chi la democrazia non sopporta e lo si fa colpendo coloro che in essa operano. Nessuno è perfetto, Presidente. Io penso che nessuno sia perfetto, ma molti di noi

con il massimo della buona volontà. E sono convinto che questo provvedimento, con le opportune modifiche che sono state proposte, possa corrispondere al meglio a questo nostro bisogno. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare i componenti della Commissione e il Presidente per l'ottimo lavoro svolto e poi mi sembra doveroso ricordare un siciliano che, in questi giorni, ha subito un gravissimo attentato. Si tratta del presidente del Parco dei Nebrodi, dottor Antoci,

meno soli. La proposta di legge oggi al nostro esame è il risultato della volontà politica di dare un seguito ai risultati a cui è pervenuta la Commissione di inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali.

Il Parlamento si è dimostrato vicino ai bisogni di ascolto e protezione di tutti coloro che contribuiscono ad amministrare la cosa pubblica negli enti locali, anche considerando tutti gli atti di sindacato ispettivo presentati da deputati e senatori, che sollecitano spiegazioni e richiedono assistenza per sindaci e amministratori locali colpiti da minacce o ritorsioni. Queste interrogazioni e interpellanze costituiscono altrettante testimonianze di come i rappresentanti della Nazione non intendano trascurare i pericolosi episodi che spesso coinvolgono gli amministratori locali, in contesti dove il rapporto tra Stato e cittadini è più diretto e meno filtrato, e dove possono manifestarsi tentativi di influenza indebita, intimidazioni e violenze. Certamente le iniziative dei parlamentari e il lavoro della Commissione d'inchiesta, pur se costituiscono importantissimi segnali della vicinanza dello Stato agli amministratori in difficoltà, rappresentano solo una parte delle iniziative e degli strumenti utili ad affrontare concretamente il problema. Tali strumenti, quindi, sono stati messi nero su bianco dal disegno di legge che oggi esaminiamo. Il testo licenziato dalla Commissione giustizia, infatti, inasprisce le sanzioni per chi commette atti di intimidazione nei confronti di chi amministra la cosa pubblica con dedizione e rispetto della legge. Le soluzioni di carattere legislativo proposte dalla Commissione hanno come scopo la realizzazione della più adeguata prevenzione e del più efficace contrasto delle intimidazioni: in questo modo si potrà assicurare un esercizio delle funzioni degli enti e degli amministratori locali libero ed efficiente. In particolare, relativamente all'articolo 338 del codice penale (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), il provvedimento estende l'applicazione della norma, da un lato, agli atti di intimidazione nei confronti dell'organo politico, amministrativo, giudiziario o dei suoi singoli componenti e, dall'altro, ai casi in cui essi sono finalizzati a: «ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Per tali fattispecie si rende pertanto possibile il ricorso alle misure cautelari e alle intercettazioni. Inoltre, con l'articolo 2 viene estesa l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza anche al predetto reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Ancora, con l'articolo 3 del disegno di legge viene inserito nel codice penale il nuovo articolo 339*-bis* relativo a nuove circostanze aggravanti: in aggiunta alle aggravanti già previste la norma prevede un'ulteriore aggravante delle pene (da un terzo alla metà) se gli atti di intimidazione (lesione, diffamazione, violenza privata, minaccia, danneggiamento) sono commessi ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. Infine, l'articolo 4 del disegno di legge modifica il testo unico sulle elezioni degli organi comunali (il decreto del introducendo un nuovo comma all'articolo 90, relativo agli atti di intimidazione nei confronti dei candidati alle elezioni: al fine di garantire una tutela specifica anche per gli aspiranti amministratori locali, si estendono le sanzioni previste per la turbativa del diritto di voto anche a coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative. Si tratta di un provvedimento largamente condiviso tra le forze politiche, che rafforza con decisione l'apparato sanzionatorio e si inserisce in una linea politica chiara e univoca portata avanti anche dal Governo. Per concludere, infatti, sembra utile ricordare che il Ministero dell'interno ha costituito l'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali che, anche attraverso delle sezioni provinciali, analizza le denunce presentate in materia, indaga sulle cause più ricorrenti di tali fenomeni e promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema della legalità dedicate soprattutto ai giovani.

siamo qui a discutere il disegno di legge scaturito dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Diciamocelo: normalmente le Commissioni d'inchiesta non danno seguito ad azioni in questo caso così non è stato e spero che tale lavoro non venga successivamente reso vano dalle dinamiche politiche delle aule parlamentari. Entrando nel merito del lavoro svolto, devo dire che durante i dodici mesi di attività i commissari hanno avuto modo, in un clima di totale condivisione, di poter analizzare un fenomeno troppo spesso

Alla base del fenomeno (escludendo volutamente le cause derivanti dalla malavita organizzata, trattate in altre sedi) vi sono cause diverse, che vanno dalle cattive aspettative degli elettori alle maldestre dichiarazioni dei candidati e poi degli eletti ad amministrare i Comuni, dalla crisi economica dilagante che colpisce sempre di più la popolazione alle rivalse personali, a volte per eccessiva concorrenza o animosità nella competizione elettorale. elettorale. Una parte della problematica è da attribuirsi all'errore interpretativo della funzione pubblica dell'amministratore. I cittadini si sentono autorizzati a pretendere trattamenti di favore o comunque eccezioni personalizzate per problemi personali che necessiterebbero di lunghi percorsi autorizzativi o comunque di modifiche dei piani programmatici dell'amministrazione, spesso accompagnati dal binomio promessa elettorale-voto. In questi casi il problema si risolverebbe con un maggiore livello di educazione civica insegnata dalle scuole primarie, che permetta almeno di comprendere che nulla può essere lasciato alla libera interpretazione delle norme da parte degli amministratori, ma tutto deve sottostare comunque a regole Ho parlato di maggiore educazione civica, anche se temo che ormai non venga più assolutamente affrontata e, quindi, bisognerebbe di nuovo gettare le basi perché nei programmi ministeriali si inizi di nuovo a parlare del ruolo di cittadino, di gestione della *res publica* e quant'altro. Per quanto riguarda poi i candidati e i loro atteggiamenti in campagna elettorale che possano dare adito a successive ritorsioni da parte degli elettori buggerati dalle false promesse, poco rimane da dire se non che i candidati ad amministrare cariche amministrative dovrebbero avere comportamenti integerrimi e non cercare con ogni mezzo il raggiungimento dei propri obiettivi. Purtroppo sappiamo che anche in questa tornata elettorale ci sono state foto di schede segnate e tutta una sequenza di avvenimenti che non mi fanno ben sperare sul futuro. Quel tipo di promessa elettorale non porta a nulla di buono e potrebbe essere limitata con una minima preselezione. Non dico di fare come ci comportiamo noi, che evitiamo candidature senza produzione di certificati penali per carichi pendenti, ma almeno prevedere informazioni preventive che potrebbero essere veicolate attraverso pubblicazioni semplici da parte del Ministero, distribuite al momento della accettazione della candidatura, che riportino doveri e diritti delle funzioni delle cariche elettive a cui ci si sta candidando. Oppure si potrebbero introdurre alcune modifiche alla legge sulla campagna elettorale per introdurre dei paletti entro i quali un candidato si possa muovere o mettendolo in guardia sulle false promesse e e sulle conseguenze di una propaganda di basso livello, magari basata il più delle volte sull'ignoranza delle norme o su opportunità politiche. Per quanto riguarda invece la situazione economica attuale, sicuramente la quotidianità è segnata da carenze di sicurezza circa la sopravvivenza economica della propria famiglia. La ricerca di un posto di lavoro stabile che possa permettere una degna esistenza ai componenti del nucleo familiare impegna molta parte della giornata e, in certi casi, la carenza di soluzioni a breve porta porta a uno scoramento dei cittadini che, a un certo punto, non sanno più dove sbattere la testa. Purtroppo la situazione fuori da queste Aule dorate ora è questa e spesso l'amministratore si trova a dover intervenire di tasca propria per alleviare le problematiche economiche dei propri cittadini. Non sempre riesce a intervenire e in breve passa, nei pensieri di chi ha un problema, dalla condizione di salvatore a quella di carnefice. L'amministratore locale è, infatti, sempre più la prima linea dello Stato, il primo e spesso il solo contatto Stato-cittadino. E gli organi centrali, giocando su questo scudo, lasciano gli amministratori locali soli, abbandonati a loro stessi, caricandoli di oneri che spesso esulano dai compiti

una migliore programmazione delle politiche governative, un aiuto da parte dello Stato che permetta magari il superamento di questo periodo di crisi dei cittadini, come ad esempio il reddito di cittadinanza ma ormai non lo diciamo più. In linea In linea generale, probabilmente una parte delle colpe deriva sempre dalla più incombente delega da parte del Governo alle prerogative coercitive nei confronti dei cittadini. Sempre più spesso, infatti, assistiamo a un Governo che non riesce a pretendere in prima persona la riscossione delle tasse o il rispetto delle regole e, dopo aver approvato univocamente tagli orizzontali alle amministrazioni locali, ha di fatto delegato a queste ultime funzioni proprie dell'organizzazione centrale, calando su di esso un ruolo meramente da esattori, senza potere decisionale e soprattutto senza portafoglio o mezzi per poter operare. questo indubbiamente provoca un innalzamento della tensione tra le parti (ovvero cittadino e amministratore locale) e contribuisce a non metterli in condizione di proteggersi da situazioni potenzialmente pericolose. Anche in questo caso sarebbe utile un incremento della coscienza civica e un riequilibrio delle aspettative, degli obblighi e delle necessità delle parti in causa, oltre che una netta distinzione di quanto di quanto il cittadino versa in tasse all'amministrazione centrale e quanto a quella locale (dalla quale si aspetta un ritorno sul territorio in servizi). Considerando che la maggior parte di coloro che sono seduti in queste Aule

ma torniamo a oggi. Gli amministratori locali si aspettano misure concrete e non solo ed esclusivamente delle pezze per garantire loro sicurezza. Si aspettano politiche generali di benessere per i territori che devono amministrare, oltre che l'allentamento di quei patti e di quelle scellerate politiche economiche italiane che strozzano i Comuni per poi soggiogarli a scelte scellerate calate dall'alto in cambio di diritti e servizi essenziali che dovrebbero essere garantiti dalla Carta, ma lasciamo all'ordine del giorno vuole essere una possibile risposta a queste esigenze, non già un ulteriore «scudo» per la casta politica, ma un sostegno per gli amministratori locali e solo per loro, anche come segno tangibile di riconoscimento di un ruolo, quello dell'amministratore locale, come prima e più importante presenza delle istituzioni nella sfera politico-amministrativa del Paese. La democrazia, come diciamo noi, comincia sempre dal basso, dai Comuni. Facciamo in modo che possa attuarsi senza violenza, né per le persone, né per le cose.

una proposta concreta. Noi abbiamo lavorato, ci siamo presi un impegno e oggi siamo in Aula per rispettarlo. Le cose venute alla luce dopo le iniziative, i vari sopralluoghi e gli incontri che abbiamo compiuto, al di là delle diversità, mostravano degli aspetti comuni: la fattispecie, quali sono gli ambiti e gli argomenti che sono spesso oggetto e a rischio di intimidazione. Penso alle cave, ai rifiuti, alle licenze commerciali, al gioco d'azzardo. Ma soprattutto gli elementi comuni che ci hanno permesso di avvertire dette esigenze e di scrivere questo disegno di legge sono stati

della previsione della punibilità di chi compie un'intimidazione sul singolo amministratore e non sul corpo collegiale ci ha spinto ad arrivare in Aula con il disegno di legge

Vorrei che mi si dica che ho avuto il privilegio di fare un percorso utile, senza mai lasciare soli gli amministratori. Vorrei che mi si riconosca - questo sì - il privilegio di partecipare a questa marcia

a maggioranza, a opposizioni e a chi utilizza le strumentalizzazioni. Abbiamo bisogno di uno Stato forte e autorevole e di amministratori che si sentano aiutati e sostenuti soprattutto ora, in un momento in cui la crisi e le difficoltà consegnano loro una responsabilità maggiore. Mi riferisco soprattutto a coloro che

L'interrogazione riguarda i tirocini nel settore della giustizia, avviati nel 2010 dalla Provincia di Roma, grazie allo stanziamento di fondi propri. Questi provvedimenti erano rivolti a cassintegrati o percettori di ammortizzatori sociali in deroga, disoccupati e inoccupati, allo scopo di smaltire l'arretrato nella giustizia civile e penale. Nel 2011 questi programmi furono presi in carico dalla Regione Lazio; nel 2012 molte Regioni decisero di effettuare gli stessi progetti; nel 2013 gli stessi furono presi in carico dal Ministero della giustizia; nel 2014 i progetti furono prorogati con la legge di stabilità. Nel corso degli anni le persone occupate si sono ridotte da 4.500 a 2.600 unità. A novembre del 2015 è stato pubblicato un bando per 1.502 tirocinanti, per una borsa di studio di dodici mesi, da inserire nel costituendo ufficio del processo, con posti distribuiti nei vari distretti giudiziari d'Italia. Tale bando ha evidenziato forti penalizzazione per la Calabria, con la previsione di soli 23 posti, per un totale di 670 aventi diritto. Dei 1.502 posti messi a bando, ne sono rimasti scoperti circa 350 in vari distretti giudiziari. Vorrei sapere, dunque, se è intenzione del Ministro assegnare i posti vacanti alla Calabria, vista la penalizzazione già subita. **Mozioni,